dei Ministri*: «Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno

ha rimodulato il calendario dei lavori alla luce dell'esigenza, rappresentata dal Presidente della 5a Commissione, di posticipare l'inizio dei lavori in Assemblea del disegno di legge di bilancio. La discussione del provvedimento in Assemblea avrà quindi inizio, ove concluso dalla Commissione, giovedì 20, alle ore 17, per proseguire - come già previsto - nelle sedute di venerdì 21 e sabato 22 dicembre, se necessario, dalle ore 9,30 senza orario di chiusura.

però io ci terrei a condividere con l'Assemblea le considerazioni che sono state fatte, considerazioni assolutamente equanimi da parte nostra. Le opposizioni hanno manifestato un disagio profondo, basato soprattutto sul fatto che fino ad ora la Commissione bilancio convocata e sconvocata nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e anche oggi. Le opposizioni hanno dimostrato una assoluta disponibilità. Non hanno esercitato attività ostruzionistiche. Hanno collaborato, naturalmente nella diversità e, a volte, nella opposizione delle rispettive posizioni politiche,

riuscisse ad arrivare a destinazione. Tuttavia, signor Presidente, non dimentichiamo - ed è quello che abbiamo comunicato al Governo e al presidente Pesco, che ringraziamo per la sua disponibilità - che se la manovra non è qui, non è ancora qui, ma è solamente un prodotto virtuale, questo non dipende dalle opposizioni. Le opposizioni hanno più volte ripetuto che quello che si è letto in questi giorni e che si è ascoltato nei telegiornali, cioè la possibile riduzione del PIL, la riduzione del rapporto *deficit*-PIL per gli anni 2019 e seguenti

sulla scorta di periodi ipotetici che ci vengono serviti dal Governo, periodi ipotetici perlopiù dell'irrealtà, perché quello che ci viene detto e ci viene promesso il giorno prima per il giorno dopo, il giorno dopo non si realizza. quindi fatto due richieste, che io ribadisco con forza. Naturalmente, ciascuno dei colleghi dell'opposizione parlerà *pro domo* propria, ma due sono sono le richieste imprescindibili alle quali vincoliamo la prosecuzione della nostra leale e disponibile collaborazione, pur se nel nostro ruolo di opposizione, con il Governo, così in Commissione come in Assemblea. chiediamo che in Commissione venga audito il ministro Tria. Noi ci troviamo ad avere un *set* di emendamenti dei relatori e un *set* di emendamenti del Governo che rappresentano solamente una minima parte del contenuto di una manovra la cui variazione sarà nell'ordine di sei, sette miliardi. Questi emendamenti, che noi abbiamo, in maniera *naif*, definito frattaglie rispetto al *core business* e al significato profondo della manovra, hanno però anch'essi anch'essi un valore economico e devono trovare anch'essi un appostamento di bilancio. Non è quindi possibile, signor Presidente, colleghi, maggioranza, signor Presidente della

cioè, si spenderà, come, dove e da parte di chi, con numeri, colleghi, maggioranza, opposizioni, finalmente chiari, esatti e che siano in grado di passare la prova della verifica della Ragioneria generale dello Stato. Questo è, in sintesi, il messaggio che noi abbiamo trasferito in Conferenza dei Capigruppo. Ci è stato proposto dal Governo un termine Ci è stato proposto dal Governo un termine del tutto virtuale, sempre in quel *trend* di periodi ipotetici che diventano dell'irrealtà e che ormai, per noi, sono realmente e concretamente inaccettabili. Ci è stato detto: si andrà in Aula giovedì alle ore 17, salvo, naturalmente, che non sia ancora terminato l'esame del provvedimento in Commissione. Noi, signor Presidente, abbiamo detto no e abbiamo votato contro questo calendario perché chiediamo, al Governo e alla maggioranza, serietà: non per il Parlamento, non solo per il Parlamento, ma soprattutto per il Paese, che sta perdendo danaro e opportunità a seguito di questa grande e inutile incertezza.*(Applausi

È inaccettabile perché alla Commissione è stato impedito di lavorare, in questi giorni: le votazioni dovevano cominciare sabato 15 dicembre e si è impedito ai parlamentari di svolgere il proprio dovere, di approfondire i temi all'interno della manovra. E perché è successo tutto questo? È successo tutto questo perché si ama parlare della manovra: la maggioranza e il Governo amano parlare della manovra, ma amano farlo fuori da questa che è l'Aula preposta per affrontare questi temi.

abbiamo chiesto la presenza del ministro Tria: evidentemente non ci vuole mettere la faccia; con tutta evidenza si sta vergognando di cosa sta succedendo a Bruxelles. Evidentemente le continue marce indietro di questa maggioranza sugli impegni che avevano preso di fronte agli italiani, che non vengono costantemente e sempre più pesantemente pesantemente rispettati, lo mettono in imbarazzo. Altrettanto si può dire del presidente Conte: abbiamo chiesto che venisse a riferire in Assemblea al più presto per farci un quadro generale sullo stato della trattativa con la Commissione europea, sui passi indietro che il nostro Governo ha dovuto fare. Invece, niente, non riceviamo mai disponibilità. Qualche settimana fa abbiamo chiesto al ministro Di Maio di venire a riferire sugli affarucci di famiglia; ci hanno detto che poi ci darà una data, e non ne sappiamo più nulla. Sperano che ce ne si dimentichi. No, signor ministro Di Maio, non ce ne dimenticheremo, così come non ci dimentichiamo di quello che sta succedendo in queste ore. Si sta cercando di fare una manovra extraparlamentare senza coinvolgere le forze politiche, senza avere un dibattito profondo all'interno della Commissione, così come era stato promesso dalla maggioranza. All'ultima Conferenza dei Capigruppo abbiamo dettato e concordato con la maggioranza regole precise; perché non vengano rispettate in maniera metodica. Il Governo e la maggioranza abbiano il coraggio di venire ad affrontare i provvedimenti che stanno presentando; o forse non li conoscono neanche loro, continuano a navigare nel buio,

Poi, una volta presentato il maxiemendamento, chiediamo di avere il tempo per subemendarlo e il tempo, nei prossimi giorni, per dibattere la manovra in Commissione. Siamo disponibili a venire a lavorare il 26 per votare questa manovra in approfondimenti, in maniera adeguata. L'assenza e l'indisponibilità del ministro Tria e del presidente Conte ci porteranno a gesti dimostrativi in Aula; quindi, il Gruppo Partito Democratico annuncia - mi auguro insieme ad altre forze dell'opposizione - di occupare questa Aula per due ore, dopo la conclusione dei lavori, per dimostrare al Governo e alla maggioranza che non si può trattare il Senato e il Parlamento in questo modo vergognoso. Marcucci, anche se normalmente i gesti rivoluzionari non si annunziano istituzionalmente; ma comunque va bene ugualmente.

abbiamo avuto continue notizie contrastanti, fughe di notizie, anticipazioni, agenzie, senza mai avere un elemento di chiarezza per capire come sta procedendo il negoziato né quali sono gli elementi su cui si sta reimpostando

che comunque si limiterà solo e unicamente alle due misure principali, quota 100 e reddito di cittadinanza. Abbiamo letto e continuiamo a leggere tutto e il contrario di tutto. Che cosa abbiamo abbiamo chiesto di strano, dopo che per giorni abbiamo dato - il presidente Pesco lo sa - tutta la nostra collaborazione? Anzi, abbiamo sollecitato l'anticipo della discussione su alcuni elementi elementi assolutamente fondamentali: ognuno di noi ha indicato elementi importanti su cui era possibile, non solo avviare il confronto, ma già cominciare a predisporre

unica preoccupazione - lo sapete perfettamente - è quella di non far rischiare al Paese anche l'esercizio provvisorio, per questo non riusciamo a comprendere perché non si vuol far in modo che ci sia un'informativa e che il Parlamento sia messo al corrente. Tutto ciò rappresenterebbe anche per voi e per il Paese un elemento

del Parlamento le difendo sempre, non soltanto quando si sta all'opposizione, ma anche quando si diventa maggioranza

innanzitutto credo si debba partire da un dato: il Governo ha presentato una manovra che ha già affrontato una lettura alla Camera, autorizzata nei saldi dalle Aule parlamentari come da prassi;

È indubbio che c'è un'interlocuzione con l'Europa nata quando è stata presentata la manovra e tale interlocuzione sta portando a delle modifiche di cui ovviamente la Commissione avrà notizia appena avrà termine. È un po' difficile chiedere, nel corso delle trattative, al Ministro dell'economia e delle finanze di venire in Commissione. Per favore, fate proseguire il collega. Gli altri hanno parlato in assoluta tranquillità. PATUANELLI

costruttivo, partendo dalle loro posizioni politiche, ma senza mai voler incrudire il rapporto e, anzi, mostrandosi sempre inclini al dialogo sulle modalità con cui si arriverà in Assemblea con la manovra. Riteniamo che proporre un calendario che preveda,

Signor Presidente, intervengo per ribadire il fatto che - lo diciamo a tutti i membri della minoranza - da parte del Governo c'è stato fin da subito un atteggiamento di profonda di profonda collaborazione, di rispetto e di volontà di approfondire e trattare i temi che la minoranza ha portato all'attenzione del Governo con alcuni emendamenti, tant'è vero che è stato chiesto anche a voi di evidenziarne alcuni. C'è una trattativa anche su tali questioni, che possono essere considerate meno importanti, ma che sono pur sempre richieste che provengono dalla minoranza. Il fatto che si sia andati lunghi con i tempi è dettato semplicemente da una ragione, sempre richiesta dalla minoranza. Mi riferisco al fatto che questo emendamento di modifica dei saldi venga esaminato in Commissione e non in Assemblea. Questo è quanto ci avete chiesto. È evidente che, nel momento in cui la trattativa sarà finita e sarà pronto l'emendamento, arriviamo in Commissione. C'è stata piena disponibilità della

a darvi il tempo necessario per poter esaminare l'emendamento sulla modifica dei saldi. Con il calendario è stato detto: se riusciamo a fare in tempo entro mercoledì sera o giovedì mattina, giovedì pomeriggio alle ore 17 iniziamo l'Aula;

mio Gruppo - hanno avuto un atteggiamento istituzionale, collaborativo e leale di fronte alla trattativa così complessa di questi giorni. nell'approvazione dei documenti di bilancio non è assolutamente responsabilità delle opposizioni, ma di una trattativa che si prolunga per colpa del Governo e di chi lo sostiene da giorni e giorni. Attendiamo da giorni in Commissione di sapere quali sono i contenuti reali di questa manovra, non i dettagli

e prioritario è ribadire che il Senato ha il diritto, oserei dire il dovere, di valutare, di giudicare e di emendare i documenti di bilancio e di farlo con tempo congruo, perché altrimenti si tratta di una beffa, di una presa in giro e credo che il Senato non abbia bisogno di essere offeso o raggirato. Per quanto ci riguarda, signor Presidente, colleghi, noi siamo disponibili a venire in Senato, tutti i giorni in cui la maggioranza lo deciderà, per svolgere una discussione corretta e approfondita sulla manovra bilancio. Il nostro obiettivo non è, da opposizione sfasciacarrozze, l'esercizio provvisorio, ma è semplicemente l'esercizio del nostro diritto-dovere di controllo e di verifica.

tra il Governo italiano e la Commissione europea è stato raggiunto e non ho motivo di dubitare che il Sottosegretario dia informazioni non corrette al Senato. Mi domando, quindi, e soprattutto domando ai colleghi dell'opposizione, se l'accordo è raggiunto,

per poi dirci venerdì mattina che il maxiemendamento si presenta al Senato e la festa è finita così. Questa sarebbe un'offesa, non solo per noi dell'opposizione, ma credo anche per i colleghi della maggioranza, che ho il sospetto che conoscano i contenuti

Per quanto riguarda invece le richieste dell'opposizione, assolutamente condivisibili, esiste in questo momento un'importante interlocuzione - credo che ne siamo tutti consapevoli - tra il Governo italiano e Bruxelles, quindi l'Unione europea e la Commissione europea.

Le richieste di poter proseguire con un'informazione compiuta da parte di tutti i parlamentari che sono intervenuti sono richieste che condivido anch'io personalmente. Credo che la Commissione non possa proseguire senza che ci sia un chiarimento dell'esito di questa interlocuzione. Mi preme però dirvi alcune tempistiche, che non possiamo ignorare. Domani mattina alle 9 si convocherà una riunione dei commissari europei e, molto probabilmente, solo in quella sede ci sarà una formalizzazione del parere della Commissione sulla proposta del Governo italiano in merito alla manovra e quindi alla possibilità di evitare la procedura di infrazione. Ovviamente dovremo attendere tutti quel momento, senza necessariamente svelare o rivelare qual è stata l'interlocuzione, perché altrimenti non ci sarebbe una possibilità di confronto e una decisione ponderata da parte della Commissione. Vi chiedo e chiedo al Governo di poter riferire in Commissione o in Aula, nel momento in cui pervenga al Governo un qualsiasi tipo di informativa in merito, e di comunicare, probabilmente solo a seguito invece di questa riunione a Bruxelles, dell'avvenuta lettera che dovrà inviare la Commissione al Parlamento italiano. la disponibilità del Presidente del Consiglio e del ministro Tria è quella di venire immediatamente a riferire a tutti voi, per garantire la centralità del Parlamento e la possibilità di proseguire i lavori in maniera ordinata su una materia così importante come la manovra, una volta che la Commissione europea abbia comunicato la sua posizione nei confronti della proposta del Governo italiano. C'è massima disponibilità da parte del Governo

adesso i presentatori della richiesta mi dicano, in un minuto di tempo, se intendono reiterare la richiesta di una votazione o se la dichiarazione del Ministro di aver accettato e assicurato che il Presidente del Consiglio verrà in Aula non appena ci sarà il pronunciamento della Commissione europea faccia venir meno la necessità di una votazione.

*(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto è stato lei a precisare che, qualora l'intervento del Ministro fosse stato denso di significato, avrebbe riaperto il dibattito. Ovviamente io prendo atto delle sue parole e mi comporto di conseguenza. Detto ciò, signor Ministro, lei non si deve scusare. Anzi, noi la ringraziamo per la testimonianza data su questa tragedia; il nostro era un applauso sincero in termini istituzionali per quello che ha fatto. Del resto, era autorevolmente rappresentato dal suo Sottosegretario, che però, signor Ministro, ha detto delle cose molto precise e - devo dire - anche reiterate in più di un'occasione. Egli ha detto che questa trattativa era conclusa e che l'emendamento che voi chiamate mini

Signor Ministro, si rende conto di cosa ci sta dicendo? Lei sta dicendo che, finché non hanno l'autorizzazione, il ministro Tria e il presidente Conte non possono venire in Aula a parlare della manovra.

il ministro Fraccaro ci è venuto a spiegare che aspettiamo per domani la decisione della Commissione europea e che vi sarà poi la disponibilità del presidente

anche un'attenta valutazione sull'ammissibilità di questi emendamenti come da Regolamento del Senato della Repubblica.

Conferenza dei Presidenti di Gruppo e credo che questo sia un buon segnale dell'efficienza di questa istituzione.

*(PD)*. Signor Presidente, prendo atto della disponibilità data dal Presidente del Consiglio: credo che sia assolutamente necessario e indispensabile, affinché il Parlamento e il Senato della Repubblica tornino al centro dell'azione relativa alla manovra di Governo. Mi auguro che la relazione che il Presidente del Consiglio domani svolgerà sia puntuale e informativa di tutti gli aspetti riguardanti la manovra.

Non sarebbe stato possibile fare altrimenti; non avremmo potuto proseguire. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: la manovra deve avere un perimetro definito, le somme di cui si sta discutendo, in una trattativa che purtroppo non ci riguarda e che si sta svolgendo al di fuori di queste Aule parlamentari, troppo ingenti e troppo cospicue per non essere oggetto di uno stop del Parlamento. Stiamo parlando di sei, sette miliardi, che non potrebbero non riflettersi sul lavoro attuale di un Parlamento che non sarebbe in grado di esaminare il quadro di insieme. Per questo riteniamo indispensabile che il Presidente del Consiglio venga a dirci qualcosa di significativo, quali sono stati i parametri del negoziato e quali saranno gli elementi di cui potremmo disporre quando tratteremo questa legge di bilancio. Soprattutto ci aspettiamo, così come ci è stato promesso (lo ripeto, il Governo ha dato la sua disponibilità e noi abbiamo, da opposizioni responsabili quali siamo, contraccambiato senza atteggiamenti ostruzionistici), che che il Governo, nel momento in cui nella persona del Presidente del Consiglio definirà il perimetro della manovra, ci dia il tempo necessario e qualcosa di più che sufficiente per poter fare sentire la nostra voce di opposizioni e presentare emendamenti in tempi congrui. Questo lo stiamo dicendo da una settimana; è molto importante che alla disponibilità dei contenuti corrisponda anche la disponibilità relativa all'attività democratica di questo Parlamento.

il presidente Conte riferirà domani in Aula. Sono soprattutto contento che il Governo abbia accettato e abbia capito che era necessario sospendere i lavori della 5a Commissione fino

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso non portare in quest'Aula oggi la richiesta di aiuto e l'urlo di dolore che arriva da 4.500 lavoratori, che stanno protestando da ieri in Calabria (a Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Lamezia e Crotone) e che rischiano di perdere il posto di lavoro il 31 dicembre. Chiedo al ministro Tria di convocare un tavolo tecnico urgente con le sigle sindacali che rappresentano i 4.500 lavoratori, ex LSU-LPU, che rischiano di perdere il posto di lavoro. È un'emergenza sociale molto importante, che va affrontata con una tempistica che non può che essere domani, perché la legge di bilancio deve prevedere quantomeno i fondi per dare un minimo di stabilità a queste famiglie. Non possiamo lasciare dei giovani ragazzi con dei genitori che non lavorano. In Calabria è impossibile trovare lavoro. Vi chiedo

Non possiamo perdere la dignità di cittadini italiani. Vi chiedo di intervenire immediatamente. Lo chiedo al ministro Tria e al presidente del Consiglio Conte.